Il Senato non è in numero legale. Senatore Belisario, se un senatore è presente in Aula e ha la tessera in mano credo sia normale e corretto che possa votare, perché non mi pare ci sia un gioco *ad excludendum*; non è che la verifica del numero legale è un modo per truccare un risultato. È vero che il risultato non cambia: il Senato non è in numero legale, dunque la seduta sarà sospesa e riprenderà tra venti minuti.

mi collego a ciò che ha testé detto il collega Legnini. Noi abbiamo stabilito in maniera dettagliata in sede di Conferenza dei Capigruppo l'ordine dei lavori, come è noto ai vertici di tutti i Gruppi (ai Presidenti o a a coloro che li rappresentavano), anche sulla base della consapevolezza unanime dell'importanza di questo disegno di legge. Tutti i Gruppi lo ritengono importante perché affronta i temi della lotta alla criminalità organizzata, della lotta alle mafie, dell'ordine pubblico nelle città, dell'immigrazione clandestina. La situazione che si è verificata non credo abbia precedenti. Se si vogliono assumere atteggiamenti di lotta politica, per carità, non mi scandalizzo di nulla; si sappia però che questo è un atteggiamento

Presidente, c'era un accordo preso nella Conferenza dei Capigruppo per procedere all'importante discussione sul disegno di legge sulla sicurezza,

Però, se andate a contare bene i voti, vedrete che nel Partito Democratico qualcuno non ve li ha dati. Dunque è inutile che vi alleiate adesso per chiedere la verifica del numero legale sull'approvazione del processo verbale quando qualcuno che vi doveva dare i voti ieri non ve li ha dati.

Voi parlate tanto, ma alla fine, quando ci sono da fare i fatti, quando ci sono da approvare le leggi che interessano i cittadini, vi interessa invece di più raccomandare gli interessi del vostro Gruppo e di chi dovete in qualche modo collocare su qualche nuova poltrona.

Fa parte della lingua italiana: chi non è italiano lo controlli sul vocabolario.

che si cerchi di ribaltare sui Gruppi di opposizione un disinteresse della maggioranza che sostiene il Governo nei confronti della discussione di questo disegno di legge. Questo è nei fatti. fatti. Noi siamo convinti della necessità di produrre leggi fatte bene, anche nelle differenze, e prova ne è che nel disegno di legge in esame vi è tutto il contributo dell'Italia dei Valori agli articoli, che sono stati in buona parte copiati, se non saccheggiati dalla maggioranza.

provvedimento legislativo non andrà fino in fondo la colpa è della maggioranza, che è tenuta a mantenere la presenza del numero legale in Aula. Noi non siamo né i vassalli né le ancelle di nessuno.

Il Senato non è in numero legale. Sospendo la seduta per venti minuti.

vorrei esprimere personalmente il mio fortissimo e profondo rammarico per il mancato svolgimento dei lavori di questa mattina che avrebbero dovuto impegnare la sola discussione generale su un tema delicatissimo qual è quello della sicurezza. Prendo atto del fatto che, nonostante in Conferenza dei Capigruppo, all'unanimità, i Gruppi avessero deciso di procedere questa mattina alla sola discussione, prevedendo anche lo sforamento delle ore 14 pur di concludere la discussione generale e di procedere la prossima settimana secondo un calendario condiviso, sul quale comunque la Conferenza dei Capigruppo si sarebbe tornata a riunire nella mattina di martedì, come facciamo sempre, che prevedeva innanzitutto un decreto-legge e poi

di procedere alla discussione generale non si effettui operazione di voto alcuna; questa è la prassi. Se vogliamo cambiare la prassi e intendere che, quando si decide che si procede alla sola discussione generale, questo comporta comunque l'esigenza di votazioni, ben venga questo cambiamento di prassi, ma è giusto ed è corretto che ciascuno, in Conferenza dei Capigruppo, d'ora in poi, si assuma le proprie responsabilità, lo dica prima, in maniera tale che i lavori d'Aula possano procedere secondo una coerenza previsionale. previsionale. Credo che sia corretto e doveroso prendere atto che, se vi sono delle esigenze e delle istanze di modificare le prassi, la Presidenza sarà sensibilissima e si adeguerà, purché tutto avvenga alla luce del sole, nella piena consapevolezza di quello che succede.

di questa importanza e rilevanza non ha avvertito la sensibilità di essere presente oggi in Aula per garantire il numero legale.

svolgimento dei lavori. Faccio altresì notare che, nella passata legislatura, l'attuale maggioranza chiedeva sistematicamente la verifica del numero legale sulla votazione del verbale anche quando c'era la discussione generale. Quindi non so a quale prassi voglia riferirsi. Ho detto prima, in sua assenza, che noi intendevamo ed intendiamo rispettare gli accordi presi in Conferenza dei Capigruppo; avvertivamo l'esigenza che su un provvedimento di tale importanza si garantisse quella presenza che la rilevanza dello stesso richiede. Solo ed esclusivamente con questo spirito, abbiamo inteso richiedere la verifica del numero legale.

il suo intervento non ci convince perché il rammarico lo dovrebbe usare anche per altre vicende che hanno interessato l'Aula nella giornata di ieri. Ma, soprattutto, non ci convince perché la sua maggioranza ha un Ministro che dichiara... che ha un Ministro che fa la guerra ai fannulloni, per cui il Parlamento deve lavorare, e lavorare sodo, non stare a casa!

Mettiamo quindi una pietra sopra questa affermazione che non aveva assolutamente nessun motivo di essere; del resto, lei ha avuto modo anche in quest'Aula di apprezzare i lavori del presidente Marini nella scorsa legislatura. Poiché sono in Aula ormai da qualche anno,

per le discussioni generali non chiedevamo - contrariamente a quanto asserito dal senatore Legnini - il numero legale. La discussione generale avveniva e PdL)* in maniera corretta, alla presenza dei senatori che intendevano essere in Aula. La scorsa legislatura ero Vice Presidente di Gruppo, ho partecipato a diversi Consigli di Presidenza e posso testimoniare che le affermazioni rese dal presidente Schifani

anche con una reazione assolutamente scomposta) cambiare una prassi, credo che voi abbiate agito contro tale prassi ed abbiate impedito, con questo atteggiamento, con la richiesta di numero legale dopo che all'unanimità la Conferenza dei Capigruppo aveva deciso di procedere oggi alla discussione generale, che il Parlamento, in particolare svolgessero correttamente e in maniera proficua una giornata di lavoro su un tema importante. Quindi, a conferma di quanto asserito onestamente poco fa dal presidente Schifani, la Lega Nord prende atto di questo atteggiamento inutilmente ostruzionistico ostruzionistico nei confronti dei lavori d'Aula e rigetta totalmente le assurde affermazioni testé rese dal presidente Belisario. Presidente, la ringrazio per la sua puntualizzazione. In realtà oggi è stata violata una prassi, perché in discussione generale e in presenza di un accordo non c'era mai stata una richiesta reiterata di numero legale sul processo verbale. Noi della maggioranza abbiamo una responsabilità, ma non è quella che dice il senatore Legnini. La nostra responsabilità è quella di esserci fidati della lealtà dell'opposizione. siamo presenti, come è possibile constatare anche ad occhio, in un numero anche doppio rispetto ai colleghi dell'opposizione. *(Applausi dai per circa 20 senatori e soltanto ricorrendo alla tecnica dei congedi, che l'opposizione conosce bene, avremmo potuto assicurare il numero legale oggi. Non l'abbiamo fatto perché non è stato mai necessario. Prendiamo atto di questa novità, una novità che segna i nostri rapporti. Il senatore Belisario potrà stare stare tranquillo: dalla settimana prossima sapremo recuperare e dimostrare di stare qui, se serve, anche per sedute notturne. Noi ci saremo tutti, come ci siamo oggi! Quello che cambierà è che non avremo più considerazione della parola data dall'altra parte! *(Vivi

a cui noi possiamo chiedere il rispetto delle prassi istituzionali. Lei, quindi, deve fare qualcosa perché la minoranza sia tutelata in un suo imprescindibile diritto;

sempre inteso dare un forte impulso all'obbligatorietà della convocazione del Parlamento in seduta comune, da un lato, e della Commissione di vigilanza RAI, dall'altro, per stimolare le forze politiche a trovare un'intesa. Sul primo punto siamo riusciti, naturalmente grazie alla buona volontà delle forze politiche che hanno poi trovato un'intesa che ha fatto convergere la maggioranza qualificata dei voti sul nuovo giudice della Corte costituzionale, ci siamo ripromessi di continuare a stimolare in maniera incessante la convocazione della Commissione di vigilanza RAI al fine di arrivare ad analogo risultato. La scelta del Presidente della Commissione di vigilanza, senatore Procacci, sfugge alla volontà dei Presidenti i quali possono, con l'azione di stimolo, esercitando quindi una *political* *suasion*, fare in modo che i partiti risolvano tale questione. Un fatto è certo, senatore Procacci: qualora la elezione del futuro Presidente della Commissione di vigilanza RAI dovesse essere individuata in un soggetto facente parte della maggioranza e non della opposizione, questo costituirebbe un fatto certamente grave sotto il profilo squisitamente politico, più che istituzionale, e meriterebbe ovviamente i doverosi commenti da parte di ciascuno di noi. Ma ciò non è avvenuto. Quello che invece oggi, senatore Procacci, la Presidenza si è permessa di ravvisare era un altro aspetto.

Non vi è dubbio che, ove necessario, questa Presidenza non si sottrarrà ad ulteriori interventi in occasione dei quali manifesterà la propria preoccupazione e cercherà, attraverso il proprio ruolo, di fare in modo che questa annosissima vicenda che si protrae da troppi, troppi anni, possa concludersi con la sottoscrizione di un sacrosanto contratto dei giornalisti i quali hanno un sacrosanto diritto.

Sono serviti cinque anni per concluderlo; adesso è concluso e siamo in presenza di una carenza di circa 870 educatori carcerari. Ho visitato personalmente alcune carceri e alcuni direttori di carceri e la Polizia penitenziaria mi hanno pregato di rivolgere al Ministro della giustizia questa interrogazione e di sollecitarla in tal senso. Anche in merito al provvedimento di cui discuteremo la settimana prossima, quello sicurezza legato anche al tema dell'immigrazione, non possiamo immaginare di assolvere al principio costituzionale della pena come forma di punizione e non anche di riabilitazione. Ci auguriamo che funzioni soprattutto la parte rieducativa. Senatrice Baio, la Presidenza è sensibilissima a questo tema e si permetterà di invitare il ministro Alfano, o in occasione di un *question time* o in occasione dell'eventuale presenza del Ministro durante il dibattito sulla sicurezza,

viaggio ufficiale all'estero, altrimenti sarei stato felicissimo di riceverli. Prego lei, eventualmente anche a mio nome, di porgere loro il mio saluto e di dare la rassicurazione che questa Presidenza si farà carico presso il Ministro della giustizia di chiedere immediata risposta.

situazione che si è creata ieri, che credo sia di una gravità estrema: mi è stata tolta la parola da parte di un Gruppo che è all'estrema destra di questo Governo e che ha intimorito i due Presidenti di

che sei andato da loro! PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, non personalizziamo il tema. Senatore Pedica, la pregherei di dare il senso della nota e di concludere il suo intervento, anche perché sto cercando di far parlare tutti per come è giusto sia, anche se dovrei chiudere la seduta. PEDICA Ieri in 580 sono stati chiamati dal tribunale e per loro tutti il pensiero era il dispiacere nei confronti dei passeggeri che si sentono inferociti, disinformati e male informati. Infatti la stampa, la stampa di regime, arringa la gente, ma non spiega anche il loro problema, che lo stipendio di un assistente di volo non è come quello dei deputati, ma è di 1.200 euro, eppure servono questa compagnia. Non sanno neanche stanno combattendo queste persone perché continuate solo a fare demagogia, non sanno dei licenziamenti e delle aberranti condizioni contrattuali che vengono Iniziano a preoccuparsi seriamente e a chiedere cosa fanno in merito le donne che siedono in Parlamento. A queste donne, se esistono in Parlamento, glielo dico io: questa assistente di volo è preoccupata perché le categorie a rischio di licenziamento sono le donne in stato interessante, quelle che hanno i figli piccoli, i portatori di handicap e chi non è in condizione di fare i turni di notte. questi assistenti e questi piloti, per essere assunti, hanno dovuto presentare il certificato del casellario giudiziale al fine di dimostrare di non avere precedenti penali, ma nessuno lo ha chiesto ai soci della CAI, a quelli che dirigeranno la compagnia, il cui casellario giudiziale è pieno di truffe allo Stato. È questo che dobbiamo denunciare!

svolgere anch'io, come hanno fatto altri, una breve riflessione sulla situazione della Commissione di vigilanza RAI. È necessario registrare - e, a questo punto, diciamo solo registrare - che, per più di 40 volte, la maggioranza ha mandato la Commissione in condizioni di assenza di numero legale, legale, con un preciso significato, espresso apertamente senza alcun infingimento: la maggioranza ha dato a intendere che voleva influire, più o meno direttamente, sulla nomina del Presidente che deve essere - per giusta consuetudine istituzionale - espresso dall'opposizione. Insomma, in parole povere, la maggioranza voleva esercitare un'influenza sul candidato dell'opposizione,

in una condizione di totale anomalia istituzionale, rappresentata dal fatto che lo stesso soggetto è il possessore dei mezzi privati di comunicazione, il titolare del potere politico e da lì, quando può, anche il controllore dei mezzi d'informazione pubblici. Questa è una cosa che purtroppo non può togliere nessuno e, quando finirà, sarà troppo tardi. Comunque, a questo punto, pur permanendo questa situazione di anomalia gravissima - che inquina alla radice

Questo da un certo punto di vista ci conforta, perché ora la Commissione ha la potestà di esprimere il Presidente. Penso che bisogna serenamente accettare il fatto che sta all'opposizione garantire la nomina del proprio candidato: è una cosa che ci si augura possa accadere nelle prossime convocazioni. Il candidato è uno solo, è di gran lunga la persona più adatta, ha la qualità e la capacità di mediazione per svolgere quel ruolo meglio di qualsiasi altro, ha una storia politica nobile alle spalle, non è affatto l'estremista che è stato indicato in modo del tutto surrettizio dai mezzi d'informazione.

dunque, ha tutti i caratteri della persona dialogante, moderata e tranquilla. sembra orientata a garantire anche nel futuro prossimo il numero legale, sta all'opposizione garantire l'elezione del proprio unico candidato.

riesca ad esprimere o meno un Presidente non lo sappiamo, ma certamente già la partecipazione è un segnale di miglioramento della situazione della trattativa politica e dell'atteggiamento dei Gruppi in relazione ai loro doveri istituzionali.

se dovessimo leggere le lettere delle centinaia di cittadini italiani che protestano contro lo sciopero dell'Alitalia sarebbero necessarie

12.600 posti di lavoro, oltre a 600 posti di tecnici degli stabilimenti di Napoli, ancora operativi. Lo si deve al lavoro intelligente del sottosegretario Letta che ha saputo mettere insieme una situazione che permette oggi all'Alitalia di volare. Quello che fa Pedica è altro: è l'istigazione allo sciopero fuori da ogni controllo. Ieri un grande quotidiano italiano riporta la foto di Pedica che sta lì a zufolare per tentare di far fare inutili scioperi, quando invece la Compagnia aerea italiana centinaia e centinaia di utenti che volano con altre linee aeree, proprio perché non hanno più la tranquillità di volare con Alitalia, grazie all'istigazione di Pedica, dei suoi amici, fatta l'altro giorno nell'aeroporto di Pedica)*. Quindi, prima di leggere queste lettere, sentiamo invece l'orgoglio di difendere quei lavoratori che stanno facendo camminare e volare l'Alitalia e quelle centinaia e centinaia di cittadini italiani che hanno dovuto cambiare linee aeree, o quei tanti cittadini stranieri che per arrivare in Italia devono trovare altre linee aeree che faranno sicuramente la ricchezza di Pedica e degli amici di Pedica.

in Aula ad inizio seduta perché impegnato in una riunione politica importante, tra l'altro su un tema lungamente dibattuto in Aula stamattina, quindi non ero presente quando il Gruppo del Partito Democratico ha richiesto una verifica del numero legale.

La questione potrebbe finire qua, se non avessi sentito dal senatore Quagliariello poco fa una denuncia di mancanza di lealtà.

slealtà avesse un significato: mi è stato riferito che la questione è stata posta in termini di coerenza da parte del Gruppo del Partito Democratico con le decisioni della Conferenza dei Capigruppo. Ora, io escludo, e lei escluderà con me, che mai nella Conferenza dei Capigruppo sia stata posta la questione del quando si sarebbe potuto esercitare il diritto di chiedere la verifica del numero legale. Tale questione non è mai stata posta, su questo punto mai è stato preso un impegno. preso un impegno. E voglio annunciare adesso formalmente in Aula che il Gruppo del Partito Democratico si riserva, ogni qualvolta lo riterrà opportuno e necessario, di chiedere la verifica del numero legale. anche dirle, Presidente, che se per caso le decisioni della Conferenza dei Capigruppo dovessero essere interpretate nel senso che la decisione all'unanimità comporta, come conseguenza, la privazione

(ne abbiamo ampia documentazione negli atti parlamentari, ma abbiamo anche documentazioni fotografiche per chi volesse prenderne visione), i comportamenti dell'opposizione nella passata legislatura, nella quale la maggioranza aveva ben altre possibilità numeriche rispetto a quelle di cui dispone la maggioranza in questa legislatura. Voglio soltanto fare questo rapido accenno per dire che mi sembra che se vogliamo

si era consolidata - dico «si era» perché evidentemente da oggi non è più così - una prassi in relazione alla quale, quando la Conferenza dei Capigruppo all'unanimità assegnava ad una seduta l'esigenza di sviluppare la discussione generale, questa decisione comportasse implicitamente, in maniera condivisa da tutti - e tale prassi è sempre stata rispettata da tutti - l'assenza di votazioni. Qualche precedente che torna alla mia memoria riguarda soltanto richieste di numero legale singole, che non si sono mai protratte nella loro entità in modo tale da impedire poi lo svolgimento della seduta.

Non sono regole scritte; ho detto soltanto che alla luce dell'evento di oggi tutti i Capigruppo e la Presidenza debbono avere per certo un fatto: questa prassi da oggi non vige più e ogni Capogruppo si deve assumere la responsabilità di sapere che anche se si decide di procedere alla discussione generale ciò non comporta l'assenza di votazioni, come invece sempre avvenuto in passato. Tutto qui: mi sono limitato a dare questo segnale, a prenderne atto. La mia amarezza nasce da questo fatto, dalla violazione di una prassi, ma è diritto dell'Aula cambiare le prassi, non è diritto della Presidenza, perché l'Aula è sovrana. La mia amarezza nasce da questo, ma è soltanto un'amarezza, perché decide l'Aula se cambiare le prassi. Le prassi per tanti anni sono state queste, collega Zanda; possono cambiare, ognuno si assumerà le proprie responsabilità, sia maggioranza che opposizione, e ognuno si adeguerà al cambiamento delle prassi. Altra amarezza deriva dal merito del tema trattato in Aula, quello di un disegno di legge ordinario sulla sicurezza per il quale si era deciso, da parte di tutti, di questa mattina, anche andando oltre le ore 14, per un'ampia discussione generale in un'estrema articolazione tra maggioranza e opposizione, trattandosi di un tema che è naturalmente caro ai cittadini e su cui i Capigruppo avevano trovato l'unanimità in ordine alla condivisione di questo percorso.

rispettivamente presidenti della Commissione ambiente e della Commissione educazione della medesima Assemblea. Invito i colleghi presenti a rivolgere loro un caloroso saluto. *(Applausi)*. È inoltre presente in tribuna una delegazione del Comune di Laives e dell'Alto Adige, che ringrazio e saluto.